Comunico che, in data 3 giugno 2008, è stato presentato il seguente disegno di legge: *dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro dell'economia e delle finanze*: «Conversione in legge del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97,

La informo che il Presidente della Repubblica con proprio decreto in data odierna, adottato su mia proposta e sentito il Consiglio dei Ministri, ha nominato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri il dott. Guido BERTOLASO, Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con decorrenza dal 23 maggio 2008. *F.to*Silvio Berlusconi».

La Conferenza dei Capigruppo, riunitasi ieri sera, ha approvato integrazioni al calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori fino al 12 giugno. Come previsto dall'ordine del giorno, questa mattina inizierà l'esame del decreto-legge recante recepimento di obblighi comunitari, che - secondo i tempi già definiti - si concluderà entro la fine della settimana, in relazione all'imminente termine di scadenza. Sempre nel corso di questa settimana sarà discusso, se concluso dalla Commissione competente, il decreto-legge sull'adeguamento delle strutture di Governo, per il quale si è proceduto alla ripartizione dei tempi tra i Gruppi. La Conferenza dei Capigruppo ha definito gli argomenti che saranno oggetto delle interrogazioni a risposta immediata (cosiddetto *question time*) previste per giovedì 5 giugno alle ore 16, vale a dire: emergenza alluvione in Piemonte e violenza sulle donne, alle quali risponderanno rispettivamente il Ministro per i rapporti con il Parlamento e il Ministro per le pari opportunità. Le scansioni dei tempi saranno le seguenti: per il primo dei predetti argomenti (alluvione in Piemonte) la Conferenza dei Capigruppo ha ritenuto di derogare eccezionalmente alla prassi consolidata. Pertanto, gli interroganti - uno per Gruppo a cominciare dai Gruppi più numerosi - avranno a disposizione 3 minuti per ciascuna domanda e 2 minuti per le repliche che seguiranno la risposta congiunta del Ministro, per 10 minuti. Per il secondo argomento (violenza sulle donne) si seguirà il consueto schema: 2 minuti per le domande; risposta congiunta del Ministro per 10 minuti; 1 minuto per le repliche. Si fa presente che la RAI metterà a disposizione un'ora di trasmissione diretta televisiva. Ove non concluso in tale ambito di tempo, il *question time* proseguirà normalmente anche al di fuori della trasmissione diretta. La prossima settimana, nelle sedute previste dal 10 al 12 giugno, oltre all'eventuale seguito del decreto-legge sull'adeguamento delle strutture di Governo, 1'Assemblea esaminerà il decreto-legge sul trasporto aereo, già approvato dal Senato, ove modificato dalla Camera dei deputati; il decreto-legge in materia di sicurezza pubblica, se concluso dalle Commissioni competenti, e la proposta di istituzione di una Commissione di inchiesta sugli infortuni sul lavoro. Per i decreti-legge sono stati ripartiti i tempi tra i Gruppi.

Signor Presidente, il decreto-legge in esame è stato emanato l'8 aprile dal Governo Prodi, in relazione ad una serie di procedure in corso presso gli organismi europei nei confronti dell'Italia per mancato adeguamento a precedenti Si tratta di una serie di adempimenti - come anche quelli contenuti negli articoli aggiuntivi introdotti nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento - in mancanza dei quali,

di ulteriore ritardo nell'applicazione delle stesse. Pertanto, le ragioni di necessità ed urgenza e l'opportunità di queste norme, nel loro insieme, sono ampiamente giustificate dagli elementi

Il compito naturalmente non è facile: queste procedure sono complesse, possono richiedere un certo periodo di tempo e, peraltro, non sono esenti da errori. Infatti, in entrambi gli articoli si prevede che non si procede al recupero di queste somme ove ricorrano entrambe le condizioni previste, e cioè gravi motivi di illegittimità della decisione di recupero, ovvero evidente errore nell'individuazione del soggetto tenuto alla restituzione dell'aiuto di Stato, nonché pericolo di un pregiudizio imminente e irreparabile per l'impresa alla quale vengono richiesti questi fondi.

Una sentenza della Corte di giustizia, infatti, aveva stabilito che l'Italia non aveva pienamente recepito la normativa europea

stabilito per il completo adeguamento delle condizioni. Queste norme sono ora inserite sostituendo il comma 6 dell'articolo 77 del decreto legislativo 3 aprile 2006, All'articolo 4 abbiamo un adeguamento alle norme europee in generale per quanto riguarda la libertà d'impresa e la libertà di stabilimento. Nella normativa italiana l'attività di recupero stragiudiziale dei crediti era ed è tuttora sottoposta ad una serie di condizioni, tra cui il fatto che l'attività possa essere esercitata soltanto

La Corte di giustizia ha rilevato che alcune di queste limitazioni sono contrarie alle normative europee. L'articolo 4, pertanto, esenta dall'affissione di queste documentazioni precedentemente previste nonché anche dall'effettivo possesso ed esercizio di sedi presso le quali affiggere queste documentazioni. Inoltre esclude i limiti territoriali per l'esercizio di questa attività, una volta ottenuta la licenza per una qualsiasi parte del territorio della Repubblica italiana. L'articolo 4-*bis*, introdotto nell'altro ramo del Parlamento, previsto in attuazione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 13 settembre 2007 in materia di concessione per la gestione di scommesse ippiche. La Corte di giustizia ha ritenuto che tale tipo di concessione vada soggetta ad una gara, ad una evidenza pubblica, che precedentemente non era prevista, e questo a tutela della libertà di stabilimento assicurata dalla normativa europea.

il riconoscimento del servizio pubblico svolto nell'ambito dell'Unione europea, quando si richiede un'esperienza professionale o una anzianità acquisita nell'esercizio di una certa attività. Con l'articolo 5 questa anzianità può essere stata conseguita anche precedentemente alle norme che riconoscevano reciprocamente tra gli Stati tra gli Stati membri dell'Unione europea tale esperienza. Pertanto, abbiamo un allargamento ed un pieno recepimento a livello comunitario della possibilità di esercitare determinati tipi di attività. All'articolo 6 6 ci sono norme riguardanti l'adeguamento di discariche di rifiuti pericolosi a determinate norme. norme. Una sentenza della Corte di giustizia aveva stabilito che le nostre norme non fossero sufficientemente precise nel determinare l'ultimazione dei lavori di adeguamento per le discariche di rifiuti pericolosi che ora viene fissato con un termine che non può essere successivo al 1° ottobre 2008. Vi sono poi norme atte a rendere pienamente operante questa previsione. L'articolo 7

una sentenza della Corte di giustizia che ci chiedeva una più stringente normativa che vietasse sbarco, trasporto e commercializzazione di esemplari di specie ittiche al di sotto della taglia minima prevista dai regolamenti comunitari e dalle norme nazionali applicabili. L'articolo

i precisi requisiti per l'esercizio delle funzioni di comandante e di primo ufficiale di coperta, a seguito del recepimento della procedura di infrazione n. 2004/2144 riguardante, per l'appunto, l'esercizio delle funzioni di comandante e di primo ufficiale di coperta.

sul luogo di lavoro e, pertanto, dà gli stessi diritti a entrambi i genitori. L'articolo 8-*quinquies* si riferisce alla composizione di organismi previsti dal decreto legislativo n. 74 del 2002. L'articolo 8-*sexies* è particolarmente rilevante perché recepisce in modo compiuto, a seguito di una procedura di infrazione, alcune norme europee riguardanti la discriminazione per qualunque motivo. In particolare, i comportamenti indesiderati che possono avere carattere discriminatorio nei confronti di determinati soggetti non devono più essere umilianti e offensivi per essere colpiti dalle sanzioni previste dalla leggi; è è sufficiente che siano umilianti od offensivi. Inoltre, viene stabilito che - su questo ci era già stata una lunga discussione all'epoca del primo recepimento

tali da fondare in termini precisi e concordanti la presunzione dell'esistenza di atti, patti o comportamenti discriminatori, spetta al convenuto l'onere di provare l'insussistenza della discriminazione.

della procedura di infrazione, che la normativa qui illustrata potesse essere introdotta, sia pure con le suddette limitazioni. Lo stesso vale per la protezione delle vittime.

L'articolo 8-*novies* riguarda una nuova disciplina per le concessioni dei diritti di uso delle radiofrequenze per la diffusione sonora e televisiva, materia peraltro oggetto della maggior parte degli emendamenti che andremo ad esaminare.

Pertanto, la Presidenza propone all'Aula di impegnare la seduta antimeridiana nella discussione generale - vi sono 13 colleghi iscritti a parlare

ricorderete, è stato oggetto, nella recente discussione alla Camera dei deputati, di una aspra contesa. Il testo, infatti, nella sua prima versione era un vero e proprio condono per le emittenti, ivi comprese quelle in posizione non propriamente legittima, e non rispondeva, nel modo più assoluto, né alla procedura di infrazione comunitaria comminata al nostro Paese nel 2005 in merito alle normative in materia e neppure alla recente sentenza della Corte di giustizia del 31 gennaio 2008. Vi è stata poi una seconda stesura e, infine, una terza, quella che oggi discutiamo.

doverosa perché, onorevoli colleghi, nel frattempo, nel passaggio dalla Camera al Senato, vi è stata una novità di cui il Governo deve tenere assolutamente conto. Mi riferisco alla recente sentenza del Consiglio di Stato che, in applicazione della citata sentenza della Corte di giustizia europea del 31 gennaio 2008,

È un punto di grande rilievo che ci riporta indietro negli anni quando, attorno al tema delle frequenze analogiche, vi fu una disputa piuttosto significativa e ci riporta ancora più indietro nel tempo quando, nel 1990, proprio in quest'Aula vi fu un atto piuttosto clamoroso, cioè l'uscita di alcuni Ministri dell'allora Governo per non approvare la cosiddetta legge Mammì; tuttora, poi, non è risolto il tema dell'attribuzione delle frequenze. È molto amara questa considerazione, nel momento in cui nel villaggio globale si discute di quale

Lawrence Lessig chiama i *creative commons*, cioè l'opportunità di utilizzare l'informazione come un bene comune; dunque, mentre questo è il tipo di dibattito che avviene in quasi tutti i Paesi evoluti e mentre questa è la normativa che ormai sta entrando in vigore pressoché in tutti i Paesi europei, noi abbiamo un buco nero di almeno 20 anni e siamo costretti ancora a discutere di un argomento che si doveva risolvere tanto tempo fa. È augurabile, quindi, che dopo la sentenza del Consiglio di Stato il Governo, riferendo alle Commissioni competenti del Parlamento, voglia finalmente mettere mano ad una *vexatissima quaestio* che altrimenti ci trasciniamo, non permettendo al nostro sistema di fare quel salto di qualità indispensabile ad un Paese maturo. È vero che il testo, nel passaggio

accezione di "licenza" a quella di "autorizzazione generale", non chiarisce pressoché nulla sui caratteri della transizione da analogico a digitale; lo stesso digitale, anche in questo testo, invece di diventare un'opportunità strategica per tutto l'universo dei *media*, appare ancora tardivamente un aggettivo di televisione, quasi che fosse una semplice attribuzione della vecchia scatola televisiva per aumentare il numero dei canali. È incerto il tempo di questo passaggio e non è chiara la necessità - che l'Europa più volte ci ha richiamato a determinare - di una non discriminazione nell'attribuzione delle nuove opportunità trasmissive. Insomma, il rischio, tutt'altro che fugato anche nella presente stesura, è che si possa perpetuare quella concentrazione televisiva che nell'analogico ha già fatto tanti danni al pluralismo e che rischia di essere moltiplicata per enne volte nel passaggio al digitale. Non c'è, dunque, equilibrio. il digitale è ancora una tecnica soprattutto a pagamento e non è ancora definita una vera strategia industriale al riguardo. Quanto al tema del reperimento delle frequenze per sopperire alle esigenze, peraltro sottolineate anche dal Consiglio di Stato, per il gruppo di Europa 7, è giusto osservare che sempre il Consiglio di Stato ha ribadito che una delle emittenti che nel 1999 non ebbe la concessione ma una mera autorizzazione a trasmettere provvisoria, cioè Retequattro, può continuare a trasmettere. Tuttavia esiste la necessità che venga fatta al più presto una verifica su tutte le frequenze eccedenti - e tante sono in Italia le doppie, triple e quadruple frequenze - e per andare incontro alle giuste esigenze di quel gruppo si effettui una verifica proprio a partire da quella che fu considerata nel nostro ordinamento un'emittente eccedente gli stessi limiti *antitrust*. Le frequenze libere sono forse poche sulla carta, ma con una ricerca più precisa si rivelano probabilmente assai maggiori di quanto si suppone. e abbiamo presentato un nostro emendamento al riguardo - che quanto prima il Governo riferisca alle Commissioni competenti sullo stato dell'arte; questa vicenda non può rimanere appesa ad un filo esile, ad una mera dichiarazione di intenti. merito, voglio aggiungere - non è vuota polemica, ma è un punto di fatto - che ci troviamo in questa situazione un po' surreale (del resto è il tema del conflitto di interessi visto da vicino), visto da vicino), e cioè che lo stesso Governo, che in qualche modo ha a che fare per via diretta con il suo Presidente del Consiglio con la materia, è lo stesso che si trova ad attribuire le frequenze ad un'emittente concorrente; non vorremmo che alla fine, in caso non si arrivasse a concludere positivamente la vertenza con l'Europa, fossero i cittadini a pagare ciò che riguarda un punto attinente alla forza

quest'Aula si appresta oggi a discutere e votare un provvedimento che ancora porta la mia firma e quella del Governo Prodi, portando a termine un lavoro che ha richiesto un grandissimo impegno per risolvere un numero notevole di infrazioni. Forse i colleghi dell'attuale maggioranza potrebbero ricordare di aver lasciato in eredità il numero record di infrazioni mai raggiunte da questo Parlamento. Avete lasciato in eredità 275 infrazioni, in parte dovute all'amministrazione centrale, molte dovute alle amministrazioni locali. Devo dire che 20 mesi di cocciutaggine, di testardaggine e di lavoro con tutte le amministrazioni

e che rappresentano un dato particolarmente importante. In particolare, lei ha già ricordato - e voglio sottolinearlo - l'inserimento delle norme sulla procedura relativa alla trasposizione delle direttive 2000/43/CE e 2000/78/CE relative alla parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica e in materia di occupazione e di condizioni di lavoro. Si tratta di un lunghissimo lavoro: avevamo cercato di inserire tali misure nel disegno di legge anti-infrazione del 16 novembre scorso, che il Parlamento non ha mai né discusso né approvato; abbiamo tentato di collocarle nella legge comunitaria, che per ragioni di tempo fu invece approvata senza modifiche; abbiamo poi provato a metterle in questo decreto-legge, ma l'ordinaria amministrazione in cui versava il Governo non ha consentito di inserire se non le sei importanti. Pertanto, ben vengano queste misure e ben venga lo sforzo che il Governo ha compiuto, recependo un lavoro fatto antecedentemente. Il punto di dissenso, però, non è solamente quello già ricordato dal collega Vita, ma è il punto relativo alla questione Autostrade. Signor rappresentante per mia parte non sono mai stata un'entusiasta della gestione Di Pietro della questione Autostrade e penso che anche nel Governo precedente una serie di pasticci siano stati certamente compiuti; mi riferisco in particolare al famoso articolo 12 risolvere questa difficoltà nel modo in cui voi avete deciso è di fatto una sanatoria, è di fatto un'accettazione per legge di convenzioni passate, presenti e future, travalicando qualunque filtro previsto per legge, sia esso il NARS, il CIPE o tutti gli altri strumenti. Insomma, siamo in presenza di una vera e propria sanatoria, che ha già suscitato non solo le nostre resistenze, ma anche prese di posizione molto critiche da parte delle Regioni. In particolare, il governatore del Veneto Galan ha già annunciato la sua contrarietà e misure contro quanto voi avete deciso di fare. Colleghi più sospettosi

con la ricerca spasmodica di imprenditori italiani che ancora né ci sono, né si manifestano, né sappiamo chi siano). Insomma, una specie di partita di giro, che, concedendo utili notevoli ad alcuni di questi imprenditori,

la questione Alitalia torna in campo, non solo perché i colleghi sono sospettosi, ma perché altrimenti non si spiega non la soluzione del problema, ma questa soluzione del problema, negoziata prima solo con Autostrade e poi estesa a tutte le altre concessionarie, in un modo in cui le verifiche sugli investimenti e sulle tariffe delle convenzioni presenti, future e persino futuribili viene accettato e decretato per legge, bypassando tutti i filtri istituzionali che il nostro regime comporta.

immettendo cose che poco c'entrano. io credo che davvero non faccia bene, a meno che non ci siano - come dicevo - retropensieri non trasparentemente dichiarati. Il tempo ci dirà, in futuro, se questi retropensieri avevano una qualche validità. Quello che è certo è che questa soluzione

perché mai abbiate voluto scegliere questa strada per risolvere un problema che indubbiamente esisteva. Per questi motivi, nell'apprezzare tutto il resto del provvedimento, esprimo un voto contrario, in particolare a partire dalla vicenda Autostrade.

Signor Presidente, colleghi senatori, rappresentanti del Governo, il decreto-legge in esame ci dà l'opportunità di svolgere ad inizio legislatura una riflessione sul modo di partecipare del nostro Paese alla costruzione del processo unitario europeo. Al di là infatti della retorica, la costruzione di un'Europa che, a mio modesto avviso, dovrà essere federale e solidale o non sarà, realizza soprattutto negli atti concreti di governo e se permettete - non per svalutare il ruolo del Governo, ma per valorizzare anche la società civile ed i poteri locali - negli atti di *governance* quotidiani. L'Italia, Paese fondatore dell'Europa e forse tra i più europeisti, ha per lunghi anni goduto di una cattiva fama per tre ragioni: la condizione del suo debito; la non rispondenza ai criteri dei fondi strutturali, con la conseguente incapacità di spesa che solo grazie al lavoro dell'allora ministro Ciampi è stata risolta a favore di tutti, a qualunque parte politica si appartenga; infine, la non rispondenza agli obblighi comunitari derivanti dai regolamenti e dalle direttive, a mano a mano approvate in sede europea. Negli anni, come ha ricordato la vice presidente Bonino, il *gap* si è ridotto, ma si è ridotto solamente dal 2006 al 2008, scendendo sotto le 200 procedure di infrazione e ricordo - per quel che poi diremo - che ciò che propone la Corte di giustizia non è qualcosa su cui riflettere, ma è immediatamente esecutivo nei Paesi dell'Unione europea, pena la procedura di infrazione ed un costo economico che paga tutta la collettività. Senonché questo decreto-legge è venuto a trovarsi, come già è stato ricordato, in una condizione politica del tutto nuova, che ha inciso sul modo in cui è stato utilizzato, fino a farlo divenire altra cosa da quello che era all'inizio. Mi preme sottolineare tale contesto, perché spero che non si ripeta in futuro, soprattutto per la legge comunitaria. Se scorriamo il testo come modificato dalla Camera, eccoci al ritorno all'effetto *band wagon* delle leggi finanziarie di un'altra epoca: alla faccia del nuovo, ci ritroviamo di fronte alle leggi di una volta, che venivano utilizzate per tutto. Nel decreto-legge sugli obblighi comunitari il Governo ha introdotto nuovi articoli di legge con un effetto *omnibus,*

delle contestazioni svolte dalla Commissione europea nella nota vicenda relativa al caso di Europa 7, ma addirittura introduce disposizioni che potrebbero rivelarsi comunitariamente illegittime e di certo non soddisfano la sostanza della sentenza resa dalla Corte di giustizia delle Comunità europee lo scorso 31 gennaio (senza ricordare la Corte costituzionale italiana e il parere del Consiglio di Stato). Questo modo di procedere non solo mette in difficoltà il nostro Paese esponendolo alla procedura di infrazione certa e al pagamento economico certo, a carico di tutta la collettività, ma, ciò che è peggio ma, ciò che è peggio dal punto di vista etico e morale, conferma, con una plastica fotografia del settore che è ormai consuetudine dalla legge Mammì alla cosiddetta controriforma Gasparri fino ai nostri giorni, l'idea che nel mondo della televisione e della comunicazione in genere vale sempre e comunque la legge del più forte, istituzionalizzando un modo di comportarsi che si ripercuote non solo a livello della vicenda Retequattro-Europa 7, ma sopratutto ai livelli inferiori, dove non esiste nemmeno la regola dell'ipocrisia buonista. Cari colleghi, in tutte le Regioni emittenti locali occupano a volte abusivamente frequenze di altri e si appropriano del diritto di altri di trasmettere; radio locali hanno impianti che superano le onde di quelle delle frequenze vicine e perfino una istituzione che dovrebbe funzionare come servizio pubblico, come Isoradio, in alcune Regioni italiane

espresso in campagna elettorale. Non solo, così agendo e senza prendere parte all'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia europea, voi operate in maniera inefficacemente conservativa anche nei confronti di chi intendete proteggere con questa decisione, togliendo a Retequattro slancio, modernità, nuova organizzazione tecnica e pubblicitaria. Trasformate un'opportunità di modernità in un peana all'antico senza fantasia, tradendo anche lo spirito imprenditoriale che era alla base di questa scelta. È un comportamento, sottosegretario Romani, comprensibile solo alla luce di una politica e di un'economia dell'eterno presente che non ha più il valore del rischio di impresa e dello spirito di iniziativa. Signora Presidente, onorevoli colleghi senatori, ho concluso. Il mio appello è affinché il Governo ritiri questo articolo proposto con emendamento oppure operi uno stralcio di esso che abbia come conseguenza l'affrontare l'argomento con nuovi e più dinamici strumenti. Come vedete, ho scientemente messo da parte il dibattito accademico sui valori per lanciare una sfida che - siamo in tema generale di obblighi comunitari - dal «Manifesto di Ventotene» ad oggi, è sulle cose concrete, sull'Europa quotidiana, sui comportamenti politici. In questa sfida oggi voi decidete ancora una volta di mostrare il vostro volto più conservatore, scettico e restio all'Europa dei cittadini e della cittadinanza attiva.

«Oggi è il momento in cui bisogna saper gettare via vecchi fardelli divenuti ingombranti, tenersi pronti al nuovo che sopraggiunge, così diverso da tutto quello che si era immaginato...». Speriamo che anche il Governo di questo Paese sia della partita.

Signor Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, signori rappresentanti del Governo,

vent'anni di questo Paese dalla legge Mammì alla legge Gasparri, ossia l'occupazione abusiva dell'etere, un bene pubblico,

un ricorso al TAR e ottenuto dalla Corte costituzionale una sentenza che è tuttora inapplicata oltre ad essere anche oggetto - lo abbiamo visto di queste sentenze con le quali la sezione sesta del Consiglio di Stato hanno respinto il ricorso in appello proposto da RTI contro Centro Europa 7 per l'annullamento della sentenza del TAR del Lazio. Insomma, i cittadini, gli utenti, quelli che pagano il canone alla RAI ricevendo spesso in cambio un'informazione non sempre oggettiva

ha quantificato in 3,5 miliardi di euro, pari a 7.000 miliardi di vecchie lire, i danni che probabilmente dovranno essere pagati.

Il ricorso di Europa 7, che puntava ad annullarne l'autorizzazione a trasmettere, viene respinto, non perché campato in aria ma perché tardivo. Qui, in un Paese dove

denunziare comportamenti che, rispetto a sentenze della Corte costituzionale e della Corte di giustizia europea,

*ad aziendam*, supererà lo scrutinio della Corte di giustizia ed anche gli altri scrutini, perché ci saranno

assegnate le frequenze ma che non può trasmettere. Sulla vicenda poi di un'altra concessione, quella di Autostrade, un monopolio naturale cui siamo abituati a fare tanti regali, ne parleranno gli altri colleghi; mi limito semplicemente ad esprimere il voto contrario dell'Italia dei Valori, perché questo è un Paese che ha bisogno di rispettare le regole del mercato e di rispettare la legalità.

*(PD)*. Signora Presidente, signori del Governo, colleghi senatori, parlerò anch'io soltanto della parte di questo provvedimento che riguarda le frequenze radiotelevisive, cioè dell'articolo

e la decisione del Governo di riformulare profondamente l'emendamento originariamente presentato ha prodotto certamente un testo più rispondente ai princìpi del diritto comunitario. L'accesa discussione alla Camera non è stata infatti il frutto di un capriccio dell'opposizione, né conteneva alcuna strumentalità politica da parte nostra, tantomeno era o poteva essere letta come espressione di una volontà di penalizzare una rete o un'azienda. Le modifiche introdotte e che oggi esaminiamo sono il minimo che si potesse fare per cominciare a rispondere in modo adeguato alle contestazioni mosse dall'Unione europea con la procedura di infrazione aperta nei confronti del nostro Paese sulle norme della cosiddetta legge Gasparri in materia di gestione delle frequenze. L'altro aspetto venuto in esame nella discussione alla Camera è stato quello relativo agli effetti della sentenza della Corte di giustizia europea del 31 gennaio scorso, intervenuta nell'ambito della controversia sull'attribuzione delle frequenze ad Europa 7. Nel testo in esame oggi vi sono riferimenti corretti al diritto comunitario; manca tuttavia un espresso riferimento a tale importante pronuncia ed in particolare al principio in essa espresso che le norme nazionali non possono (sottolineo, non possono) essere interpretate nel senso di escludere dall'assegnazione di frequenze i soggetti che ne hanno titolo. Il testo approvato dalla Camera, pur essendo, dunque, un passo in avanti considerevole, va a nostro giudizio (mi rivolgo al Governo) ulteriormente migliorato tenendo conto, tra l'altro, delle novità intervenute a seguito della sentenza del Consiglio di Stato che ha tradotto nell'ordinamento nazionale i princìpi enunciati dalla Corte di giustizia europea. Il Consiglio di Stato ha disposto, infatti, che si provveda, da parte del Governo, a rispondere ad Europa 7 sulla richiesta di assegnazione di frequenze applicando quei criteri di non discriminazione, di trasparenza e di proporzionalità sottolineati dalla Corte di giustizia europea stessa. Anche nella nostra discussione, dunque, senza alcun intento strumentale, vorremmo richiamare la necessità di integrare il testo, tenendo conto che quanto affermato dal Consiglio di Stato e, più in generale, i princìpi fondamentali dell'ordinamento comunitario di settore, vanno rispettati. In questa chiave è stato da noi presentato (lo ricordava il collega Vita: da lui, da me, da altri colleghi) un emendamento che tende a dare certezza e chiarezza al procedimento che il Governo è chiamato ad attivare a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato. Ritenendo noi in particolare che un intervento del genere sia estremamente delicato sul piano del complessivo assetto pluralistico del sistema radiotelevisivo italiano, noi pensiamo, ed invitiamo a considerare, che il Governo debba avvalersi dell'acquisizione dei pareri delle competenti Commissioni parlamentari. ultimo elemento di indicazione per un attivo impegno del Governo nel recupero delle frequenze necessarie. Nel quadro attuale esistono spazi per poter proficuamente operare al fine di assegnare le frequenze necessarie, soprattutto, ad evitare una condanna allo Stato italiano o una procedura di risarcimento che sarebbe onerosa per tutti i contribuenti. Un esito del genere non sarebbe, infatti, una cosa di cui vantarsi né per il Governo né per l'intero Parlamento. La nostra speranza è che sia possibile aprire una stagione nuova, di reale apertura del sistema radiotelevisivo, di innovazione tecnologica e di costruzione del futuro. È finito a nostro giudizio il tempo del cosiddetto generale assentimento, che non è, come sanno i giuristi, un alto ufficiale delle Forze armate, bensì la traduzione un po' burocratica dell'abitudine italiana ad approvare norme che fotografano esclusivamente l'esistente, ovvero, come direbbero a Napoli, la traduzione burocratica di un motto: «chi ha avuto ha avuto, chi ha dato ha dato, scurdammoce 'o passato». Una prassi più che decennale, nel modo di procedere politico e legislativo del nostro Paese, che a nostro giudizio non ha portato bene a nessuno. La ringrazio, signor Presidente.

dell'articolo 8-*duodecies*, che approva tutte le convenzioni già sottoscritte tra ANAS e concessionarie alla data dell'entrata in vigore del presente decreto‑legge nel testo dello schema originario firmato dalle concessionarie, evitando i passaggi e le conseguenti clausole e limitazioni imposte da Commissioni parlamentari, NARS, CIPE, associazioni di consumatori e di utenti, eccetera.

Si ritiene che l'approvazione di questo articolo potrà innescare una serie di ricorsi da parte delle società concessionarie che non hanno ancora sottoscritto con ANAS la convenzione unica alla data dell'entrata in vigore di questo decreto-legge

ai fini dell'approvazione della stessa. Si ritiene infatti che il presente articolo crei delle discriminazioni tra le società concessionarie che hanno già sottoscritto la convenzione unica con l'ANAS e quelle che invece non hanno ancora concluso gli atti. Ciò sicuramente potrebbe avere ripercussioni negative anche sui piani finanziari sullo sblocco delle opere stradali in programmazione. Tenuto conto che la data di scadenza del decreto-legge impedisce qualsiasi

in maniera analoga a quanto disposto dal comma 2, primo periodo, dell'articolo 8-*duodecies* anche le Convenzioni Uniche delle società concessionarie autostradali che, alla data dell'entrata in vigore del presente decreto-legge, non hanno ancora sottoscritto gli schemi di convenzione con ANAS S.p.a.».

come l'Italia intenda stare in Europa, con quale politica, con quale idea stessa di Europa; temi già affrontati, naturalmente molto meglio di me, nell'intervento della presidente Bonino. Come si sa, il decreto‑legge in esame, almeno nel testo precedente, vale a dire prima degli ulteriori emendamenti dell'attuale Governo (che qualcuno ha chiamato incursioni del Governo), è finalizzato alla risoluzione di procedure di infrazione per le quali il mancato adeguamento, dato il tempo trascorso e lo stato di avanzamento delle procedure stesse, porterebbe con certezza a pesanti sanzioni pecuniarie. Prima di procedere a sviluppare questo tema generale che ritengo più rilevante, vorrei richiamare anche io l'attenzione sul punto di merito riferito proprio ad una delle cosiddette incursioni, cioè all'articolo 8-*duodecies,* riguardante le concessioni autostradali, nonché le convenzioni tra ANAS e concessionarie, che così compiutamente ha già affrontato la presidente Bonino nel suo intervento con cui sono completamente d'accordo.

a presunti errori del Governo Prodi, a pasticci che questo testo si proporrebbe di rimediare.

la messa in mora: siamo certi, però, che se non provvederemo in altro senso, per i prossimi trent'anni e senza verifiche, l'attuale concessionaria si assicura aumenti tariffari garantiti, senza contropartite in termini di servizi. Qui non si tratta di cultura del sospetto,

e cioè la preoccupazione che questa formulazione possa in qualche modo pregiudicare l'avvio della Pedemontana, e mi spiego.

non ha un grande interesse a dare avvio ad una nuova realizzazione, che permetterebbe di sgravare significativamente l'attuale traffico dalle autostrade di cui è beneficiaria.

un Governo con un'alta percentuale di Ministri lombardi: tuttavia, come milanese e come lombarda, posso assicurare che non è arrivato niente al nostro territorio, dal punto di vista degli investimenti.

disattenzioni per il nostro territorio. Chiudo questa parentesi per tornare al ragionamento che mi premeva. É già stato ricordato che nel periodo 2001-2006 si è accumulato un numero tale di infrazioni in numerose materie e settori, da richiedere un particolare sforzo da parte del Governo Prodi, al quale va dato atto di un impegno che ha fatto

di Paese virtuoso, come dovrebbe essere per uno dei Paesi fondatori della Comunità europea, oggi Unione europea. Questo mi sembra il punto di interesse politico: vorrei sapere se c'è spazio in questo dibattito o almeno nella replica del Governo per capire se ci troveremo ancora, tra qualche anno, ai 300 provvedimenti, a dover ricorrere ancora a decreti per sanare le situazioni, o se invece il riferimento alla legislazione europea, europea, riconosciuta nella sua legittimità, sarà fondamento e punto di riferimento abituale per il Governo e i legislatori italiani. È questo uno sforzo comune che vogliamo fare insieme, o da parte del Governo e della maggioranza che lo sostiene c'è un orientamento politico diverso nei confronti delle politiche europee? Sembra ci siamo già dimenticati, mentre discutiamo di questo decreto, che la settimana scorsa abbiamo votato il prestito ponte verso l'ignoto per Alitalia, prima ancora che il Governo rispondesse alle obiezioni sollevate dalla Commissione europea. Il presidente Berlusconi, peraltro, in una delle sue abituali e spiritose esternazioni, sempre a proposito del prestito Alitalia, ha detto qualcosa del tipo (cito a senso)

un dibattito oggettivo e laico, come è giusto fare nel momento in cui si discute sull'assetto dell'informazione e sulla questione sulla questione frequenziale: non bisogna farne, evidentemente, una guerra di religione. Facendo riferimento agli interventi svolti da qualche collega che mi ha preceduto, credo che il Consiglio di Stato, con la sua recentissima sentenza, abbia contribuito a rasserenare il clima, dopo 9 anni di battaglie e di polemiche: Retequattro può continuare a trasmettere e, successivamente, il Governo si pronuncerà sulle rivendicazioni frequenziali di Europa 7. Questa sentenza, però, smonta l'architettura delle polemiche che sono state innescate alla Camera e ne svela anche la pretestuosità, perché questo provvedimento non ha mai nemmeno lambito lontanamente la vicenda Retequattro-Europa 7. Veniamo all'Europa. Cosa ci ha contestato il commissario Kroes? La disciplina del titolo abilitativo della licenza, che non era conforme al regime europeo dell'autorizzazione generale, l'esclusiva dell'acquisizione delle frequenze permessa unicamente agli operatori esistenti provocando una chiusura del mercato; la non definizione di un limite temporale che introducesse un nuovo regime digitale, con la conclusione dell'esercizio degli impianti analogici e la conseguente restituzione delle frequenze non utilizzate. Ora, per evitare polemiche, tralasciamo l'inerzia (a nostro avviso colpevole) del precedente Governo, che pensava di risolvere tutto con la prima legge Gentiloni riducendo il fatturato di Mediaset di circa un quarto, come se in questa materia si potesse intervenire per legge. Però questo decreto, come giustamente ha ricordato il sottosegretario Romani anche alla Camera, risponde all'Europa su tutto, tranne che sulla definizione del limite temporale, perché la seconda parte del comma 3 dell'articolo 8-*novies* (che è stato lungamente in discussione alla Camera) ha evidentemente sollecitato la fervida fantasia dei colleghi, che ne hanno chiesto la soppressione. Su questi temi c'è la tendenza a non entrare nello specifico dei provvedimenti, ma - lo abbiamo constatato - a sparare demagogicamente nel mucchio. Sono state dette tante inesattezze. Avete finto di scandalizzarvi su determinate questioni, come sulla vicenda Europa 7, inflazionata e assai poco conosciuta e controversa. Molti furono i dubbi sul disciplinare che autorizzò l'editore Di Stefano a

C'è un'emittente satellitare, sul *bouquet* di Sky, al canale 924 (che contrariamente ad altre, peraltro, non è nemmeno rilevata da Auditel), che si chiama Libera TV, Libera TV, che è l'organo ufficiale di Democrazia Europea, di cui credo D'Antoni sia l'unico rappresentante in Parlamento. Libera TV ha ottenuto finanziamenti statali nel 2005 per 700.000 euro e nel 2006 per 2.400.000 euro per 2.400.000 euro e ha già presentato, ovviamente, domanda anche per il 2007. Sia chiaro che non c'è nulla di illecito, perché è la legge n. 112 del 2004 che consente satellitari organo di partito di godere di qualche finanziamento; ho anche qualche responsabilità perché fu mio l'emendamento presentato in quella sede, ma io consideravo i partiti veri e, soprattutto, le televisioni con un palinsesto serio, i cui ascolti fossero rilevati dall'Auditel. La nostra era una proposta seria e propedeutica alla soppressione dei finanziamenti di tutti quei giornaletti che nessuno legge, nessuno compra e che sono adottati quali organi ufficiali di partiti inesistenti. inesistenti. Anche una moderna configurazione legislativa, però, é stata evidentemente disattesa. Sapete chi c'è dietro Libera TV, colleghi del centrosinistra? C'è un sistema di scatole cinesi, tutte indebitate, che fanno riferimento alla Fincentro1, che è al 98 per cento nelle mani di Francesco Di Stefano, l'imprenditore di Europa 7 così tanto idolatrato dalla sinistra. Il rovescio della medaglia riguardante questo editore non interessa la sinistra, i benefìci e i favori di cui gode evidentemente non interessano. Nelle stesse condizioni c'è anche Nessuno TV, organo di un fantomatico movimento Ulisse e sostenuto da alcuni colleghi illustri e prestigiosi del centrosinistra. Ebbene, Libera TV e Nessuno TV hanno ottenuto nel 2006 6,6 milioni di euro di provvidenze contro i poco più di 8 milioni destinati a tutto il mondo dell'emittenza locale. Sono queste le vergogne di cui vorremmo sentir parlare anche dall'altra parte dell'emiciclo. Cosa voglio dire ai colleghi del centrosinistra? Che occorre spogliarsi di ogni faziosità e parlare di sistema radiotelevisivo non solo perché l'evoluzione tecnologica in atto impone costanti aggiornamenti legislativi;

siamo interessati a disciplinare ben altre migrazioni epocali che preoccupano la Nazione. Voi vi occupate solo della migrazione di Retequattro sul satellite, ma siete stati battuti anche su questo dal Consiglio di Stato; non possiamo ragionare con i rancori legati all'analogico che tra poco sparirà. C'è chi resta ancorato al difficile tema delle frequenze - che ha attraversato trasversalmente diversi Governi di diverso colore - quando il mondo fuori già pensa *next* *generation* *network*, cioè alla trasmissione dei dati su banda larga. Noi siamo ancora al doppino di rame, mentre gli altri sono già alle fibre ottiche e corrono rapidamente sull'autostrada dello sviluppo. *generation* *network*) qualcosa come 50 miliardi dollari, che saranno in grado di aumentare il prodotto interno lordo di 1.550 miliardi di dollari. Anche sulle NGN avremo la ripetizione - colleghi, ve lo anticipo - di un caso simile a quello delle frequenze in analogico perché, come si sa, Telecom detiene l'unica rete fissa veramente nazionale, che è in rame. L'autostrada c'è, ma è sostanzialmente di Telecom. Che ne sarà degli altri operatori? La televisione viaggia sui telefonini, l'IPTV è ormai scatenata, la *Web* Tv anche e noi abbiamo bloccato il Parlamento, fraintendendo per altro il senso della norma, sulle frequenze analogiche di La Tv del futuro è *on demand*, è interattiva e noi ci balocchiamo ancora sul *jurassic* *park* dell'analogico! La questione non è la risorsa frequenziale; il futuro è dominato dalla capacità trasmissiva, dove fare televisione significa anche la proprietà degli impianti ma soprattutto la fornitura dei contenuti. È questa l'architrave su cui regge il digitale, dove abbiamo operato una distinzione tra l'operatore di rete e il fornitore di contenuti proprio per aumentare ed incentivare il pluralismo nell'informazione e questo è contenuto nella legge Gasparri, piaccia o no. onorevoli colleghi, fuori c'è una "prateria" da disciplinare. Evitiamo di stare qui a contorcerci su queste miserie, che peraltro appartengono veramente al trapassato remoto. Noi come legislatori non possiamo condividere responsabilità che inchiodano il sistema industriale, in questo caso televisivo che, se dipendesse da qualche collega del centrosinistra, probabilmente produrrebbe ancora programmi in bianco e nero. Due anni non vi sono bastati per partorire il riordino del sistema, né - e lo abbiamo colto qui in Senato

l'articolo 8-*quater* modifica, al primo comma, il codice delle pari opportunità tra uomo e donna e, al secondo, il testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità. Ci è parso giusto focalizzare con un ordine del giorno l'attenzione dell'Aula del Senato proprio su questi temi. Mi sia consentito svolgere L'obiettivo di Lisbona, ossia il raggiungimento del tasso di occupazione femminile del 60 per cento entro il 2010, sembra, a questo punto, abbastanza irraggiungibile.

La manifesta disoccupazione femminile si riflette sul tasso di occupazione dell'intera popolazione, che nel 2006 è stato del 58,4 per cento, rispetto a una media europea del 64 Tale situazione impone una strategia politico-programmatica urgente nelle politiche a favore delle donne, diretta ad innalzare l'occupazione femminile e ad equiparare le condizioni di partenza nella società tra uomini e donne. I giovani che desiderano, in piena autonomia e indipendenza, sposarsi e mettere al mondo dei figli vedono infranto questo loro desiderio di fronte a problematiche molto difficili da risolvere.

La famiglia, nonostante in questi ultimi anni abbia subito attacchi da parte di una politica tendente alla sua disgregazione, rappresenta ancora il pilastro su cui si fondano le comunità locali, il sistema educativo, le strutture di produzione e di reddito e il contenimento delle forme di disagio sociale. È necessario, quindi, mettere in campo nuovi strumenti a sostegno delle responsabilità familiari e, soprattutto, misure che ne definiscano in modo coerente il suo carattere di soggetto attivo, titolare di diritti e di doveri. Si rende in altri termini urgente e non più procrastinabile un impegno concreto nella tutela del ruolo sociale della famiglia. È doveroso garantire il diritto di ogni persona a formarsi una famiglia ad essere inserita nella comunità familiare. È altresì doveroso sostenere il diritto delle famiglie al libero svolgimento delle proprie funzioni sociali, riconoscere la rilevanza sociale e personale della maternità e della paternità, sostenendo in modo più adeguato la corresponsabilità dei genitori negli impegni di cura ed educazione

in particolar modo per i nuclei familiari con persone diversamente abili, al fine di invertire il *trend* demografico negativo che vede il nostro Paese tra i Paesi europei e mondiali con il più basso tasso di natalità».

l'apologia del pluralismo tecnologico condotta pochi minuti fa in quest'Aula non può nascondere il fatto che la situazione della comunicazione e dell'informazione in Italia ha costituito negli ultimi due decenni la malattia di fondo della democrazia italiana. Sono avvenute cose che non sono accadute in nessun'altra democrazia: per riparare o per far finta di riparare a questa malattia sono stati presi provvedimenti che in nessun'altra democrazia sarebbero stati assunti.

con il diritto comunitario una normativa nazionale la cui applicazione conduca a che un operatore titolare di una concessione si trovi nell'impossibilità di trasmettere in mancanza di frequenze di trasmissione assegnate sulla base di criteri obiettivi, trasparenti e non discriminatori». Siamo, pertanto, di fronte ad una situazione in cui nel prossimo futuro questo obbligo con assoluta sicurezza non sarà rispettato; anzi, per coprire l'obbligo non rispettato, si profila una sorta di piccolo mostro fiscale che probabilmente la voce popolare fotograferà come la «tassa su Retequattro». Noi siamo sotto il peso di un fatto compiuto, che è iniziato tanto tempo fa (almeno due decenni fa), cosiddetta legge Mammì, imposta al costo di far uscire dal Governo un congruo pacchetto di Ministri, perché bisognava ratificare un monopolio privato delle telecomunicazioni. era di per sé abbastanza scandalosa, ma era niente rispetto a quello che sarebbe avvenuto dopo, perché il titolare di questo monopolio privato delle telecomunicazioni, allora distante dalla politica, negli anni successivi sarebbe diventato di volta in volta Presidente del Consiglio o capo dell'opposizione. Si è così configurata un'anomalia istituzionale, ignota in Europa ed in qualsiasi altro Paese democratico del mondo, democratico del mondo, che non si può fotografare soltanto sotto il titolo di «conflitto di interessi». Infatti, i conflitti di interessi riguardano le persone che hanno sostanze e che si trovano a legiferare

il rapporto tra la formazione dell'opinione pubblica, il consenso elettorale e la rappresentanza politica. Che fare? Il galateo ha imposto a molti colleghi di auspicare che il Governo sappia trovare il modo di soddisfare il bisogno di frequenze della rete che finora è stata pervicacemente e costantemente esclusa dall'accesso all'uso dell'etere, se non per piccoli particolari trascurabili. È forse doveroso in quest'Aula unirsi a tale auspicio, ma il ritratto realistico della situazione ci porta a dire che invece si può avere una sostanziale diffidenza verso questa possibilità e soprattutto verso il fatto che si possa modificare alla radice un'anomalia istituzionale che rappresenta la malattia endemica della democrazia italiana. La situazione è tale per cui, quando il titolare del monopolio privato delle comunicazioni è all'opposizione, si configura un duopolio nelle telecomunicazioni; quando, invece, il titolare è al Governo si configura un monopolio o un quasi monopolio, un quasi monopolio, limitato - appunto - da questa efflorescenza lussureggiante della tecnologia moderna, che però è tutta futuribile, scarsamente attuale e in ogni caso non ha più un effetto retroattivo sull'effetto iniziale di tale anomalia. Quindi, ce la teniamo comunque, c'è ormai il peso di un fatto compiuto; tutto ciò che potrà venire d'ora in poi non modifica lo stato precedente, che rappresenta appunto la ferita della democrazia in questione. Il Gruppo Italia dei Valori di fronte a questa situazione di futuro possibile, quasi di monopolio, s'impegna a vigilare con la massima attenzione, sia sul fenomeno in generale sia sul fatto che le televisioni e le comunicazioni pubbliche non vengano sottoposte ad un imperio incontrollabile.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, è inutile ripetere quello che abbiamo già detto, cioè che la legge comunitaria dovrebbe essere la sede corretta per l'attuazione degli obblighi comunitari e che questo

La seconda procedura d'infrazione a livello comunitario, avviata dalla Commissione europea contro l'Italia, terminerà infatti tra più di un anno e, quindi, avevamo un anno di tempo per esaminare la comunicazione della Commissione europea 2007/C nella quale sono contenute le istruzioni rivolte agli Stati membri per il recupero degli aiuti di Stato considerati illegittimi dalla Commissione europea. Tuttavia, il Governo Prodi-Bonino ha adottato questo decreto-legge nell'imminenza delle elezioni, probabilmente per attribuirsi una valenza europeista, come abbiamo peraltro sentito in quest'Aula, e per evitare una futura condanna, senza però minimamente curarsi della sorte delle imprese italiane che devono restituire importi spesso considerevoli, considerati aiuti di Stato illegittimi dalla Commissione europea. Queste imprese vedono dal testo degli articoli 1 e 2 di questo decreto‑legge notevolmente limitati i propri diritti di difesa di fronte ad ingiunzioni, ruoli o cartelle esattoriali di considerevole importo. Proprio in questi giorni il tribunale di Milano nella sua sua prima sentenza di applicazione del decreto-legge considera gli articoli 1 e 2 sospetti di illegittimità costituzionale per la restrizione del diritto di difesa delle nostre imprese.

si chiede a queste imprese di restituire tali imposte non pagate considerate aiuti di Stato. In secondo luogo, le agevolazioni contributive godute dalle imprese per i contratti di formazione e lavoro; anch'esse considerate aiuti di Stato e oggi, a distanza di anni, se ne chiede la restituzione. gli sgravi contributivi per le imprese in crisi occupazionale sottoposte a procedura di amministrazione straordinaria. Sono tre casi - ma ce ne sono tanti altri - di situazioni non valutate con ponderazione nell'ambito di questo provvedimento, le concrete possibilità che hanno i giudici di sospendere i titoli di pagamento sono ormai ridotte al lumicino, se non azzerate completamente. rappresento un caso concreto per capire come a fronte di articoli che appaiono roboanti di europeismo, in realtà ci siano seri rischi di tenuta di aziende oggi esistenti nel nostro Paese, di quelle poche aziende che resistono sul nostro territorio:

nel 2003, grazie ad una legge del Parlamento italiano, ha ottenuto degli sgravi contributivi; era infatti in una situazione di crisi occupazionale e di estrema difficoltà: un decreto-legge, poi convertito in legge, concesse la possibilità a questa impresa di avere degli sgravi contributivi. Ebbene, a distanza di cinque anni si considerano quegli sgravi contributivi aiuti di Stato e s'impone a tale azienda di restituirli: stiamo parlando di 10 milioni di euro; per la precisione 9.754.000 euro, di cui 8.203.000 euro di sgravi, 1.117.000 euro di interessi e 433.000 euro di aggio di riscossione; cioè l'ESATRI per notificare una cartella esattoriale chiede 433.000 euro all'azienda. Qui si potrebbe anche essere un po' ironici: credo che degli esattori, nelle altre zone d'Italia, costino meno di 433.000 euro per notificare un pezzo di carta. Ebbene, questa impresa si era rivolta al tribunale di Brescia chiedendo la sospensione dell'esecutività di questa ingiunzione dell'agenzia di Brescia dell'INPS; il tribunale di Brescia, valutando il pericolo irreparabile derivante da quest'atto per la liquidità dell'impresa, aveva sospeso l'esecutività del provvedimento. Purtroppo questo decreto-legge ha obbligato il tribunale di Brescia a revocare la sospensione dell'esecutività; quindi l'INPS, ai primi di maggio, ha chiesto all'impresa di versare i 10 milioni di euro. euro. Noi raccomandiamo al Governo di fare ciò che non ha fatto il Governo Prodi-Bonino, cioè di dare istruzioni (almeno agli uffici periferici, all'Agenzia delle entrate, all'INPS) di valutare le situazioni critiche di recupero degli aiuti di Stato dichiarati illegittimi dalla Commissione europea, per non aggravare quelle situazioni di crisi aziendale che sono già in atto.

Ma certamente - e concludo - se diminuire le infrazioni comunitarie da 275 a 185, come ci ha detto la collega Bonino, significa distruggere un patrimonio di imprese che è stato creato negli anni, allora noi non possiamo seguire questa linea suicida. Confidiamo che il Governo non voglia perseguire questa linea e voglia invece valutare caso per caso ogni singola fattispecie, per non distruggere un patrimonio occupazionale e di imprese sino ad oggi maturato nel nostro territorio.

Sulla concessionarie autostradali a me pare che si sia fatta molta confusione: si sono tentate strumentalizzazioni, qualcuno (soprattutto alla Camera) ha parlato di "emendamento Ermolli", altri (anche la senatrice Bonino) ha fatto un retropensiero, fatto un retropensiero, dicendo che questo è un regalo che si fa ad alcune concessionarie perché parteciperanno al gruppo che interverrà nel processo di privatizzazione Io credo che, per la qualità dei nostri dibattiti, dovremmo sempre rimetterci alla realtà delle carte, ai fatti formali e concreti che stanno di fronte alle proposte che di volta in volta ci vengono avanzate. Sulla questione delle concessionarie, così com'è stato osservato in Commissione, credo che si debba fare un passo indietro e tornare a due anni fa, quando il ministro Di Pietro, censurando la storia del sistema concessorio autostradale nel nostro Paese, intervenne a gamba tesa con un decreto che azzerò tutte le convenzioni in essere; convenzioni peraltro stipulate in modo libero, corretto e trasparente da parte dei concessionari con lo Stato e, per esso, con una sua articolazione: l'ANAS. Questo provvedimento del Governo, il famigerato articolo 12 del decreto-legge n. 262 del 2006, venne contestato dall'Unione europea, che a più riprese ha ricordato al nostro Paese che, se e in quanto vuole rimanere in Europa, deve rispettare i princìpi del diritto comunitario e quindi non può fare quello che immaginava poter fare il ministro Di Pietro. A seguito di quel provvedimento sciagurato, il sistema autostradale è entrato in crisi, tanto che dal maggio 2006 ad oggi non si ricordano interventi realizzati in questo comparto strategico e importante del nostro Paese, come ha ricordato il presidente dell'AISCAT in un'audizione dello scorso anno - il sistema è collassato. Quindi avete la responsabilità storica e politica di aver creato, in questi due anni, il collasso del sistema. Sono partite tre istruttorie da parte dell'Unione europea, per iniziativa

aveva la presunzione di cancellare tutte le convenzioni in essere, ma addirittura attribuiva ai concessionari l'impegno di operare come fossero amministrazioni aggiudicatrici. Badate bene (perché la qualità delle persone e delle proposte bisogna

il ministro Di Pietro, per tentare di salvarsi in angolo cosa fa? Chiede un parere al Consiglio di Stato; saputo, di lì a poco, che il Consiglio di Stato evidentemente non può seguirlo sulla strada che lui intende perseguire, chiede allo stesso Consiglio di Stato di considerare non inviata la richiesta di parere e così finisce

per il sistema autostradale, che ha realizzato interamente senza che lo Stato italiano tirasse fuori una lira: infatti non parliamo di stanziamenti, bensì di finanziamenti che si pagano con la gestione del sistema autostradale.

questo è il contenuto vero dell'emendamento al nostro esame. Dopodiché, siamo certi che con l'approvazione di questo decreto ripartiranno gli investimenti ed il sistema autostradale, che ha accumulato ritardi decennali, potrà aggiornarsi ed adeguarsi in maniera, a mio parere, assai propria. Cosa rimane da fare dopo aver sbloccato dette convenzioni? Secondo la mia opinione occorrerà modificare il famigerato articolo 12, perché anche approvando la norma in esame rimarrà in vigore

secondo la mia opinione - lo dico sottovoce - dovremmo leggere un po' meno i giornali e affidarci di più alle carte, ai dispositivi delle sentenze del Consiglio di Stato, ai decreti, alle direttive europee, allo scambio di lettere che l'Europa ci ha inviato, ricordando che anche in questo settore dobbiamo essere più europei.

nella normativa al nostro esame: questo decreto altro non fa che recepire punto per punto i rilievi del Commissario dell'Unione europea: niente di più e niente di meno. avviso è stato frutto di strumentalizzazioni concentrare il dibattito su Retequattro perché - e lo sanno bene quelli che seguono queste vicende - essa è a posto dal 2003, cioè dall'entrata in vigore del nuovo *anti**trust* analogico digitale. Infatti, nel parere motivato del commissario Kroes non si parla di autorizzazioni al posto di licenza, ma di frequenze digitali. Quindi, non cambia nulla. L'Europa non ci ha chiesto di cambiare qualcosa in ordine alle trasmissioni o alle autorizzazioni analogiche. In questo senso, credo che noi dobbiamo rispettare le norme per quello che sono: non ci sono sanatorie di alcun tipo in questa norma, perché chi opera oggi nell'analogico continuerà ad operare Si tratta, al contrario, di norme che vogliono aprire al mercato digitale facilitando l'ingresso di nuovi operatori. Non si vuole raggirare l'Europa; anzi, ci si vuole

Berlusconi ha vinto le elezioni nel 1994 perché aveva le televisioni, Berlusconi continua ad essere protagonista della vita politica perché ha le televisioni, Berlusconi è Presidente del Consiglio o capo dell'opposizione in virtù del

Signor Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, signori rappresentanti del Governo, il provvedimento oggi in discussione e successivamente all'approvazione dell'Aula costituisce nella vita ordinaria del lavoro parlamentare una particolare eccezionalità, dovuta non solo alla natura dello strumento legislativo, proprio della decretazione d'urgenza, ma soprattutto in base alla caratteristica temporale in cui il decreto-legge è stato emanato e alla conseguente temporalità in cui la legge viene approvata. Come è noto, si tratta della conversione di un decreto-legge finalizzato a sanare una serie di infrazioni in cui il nostro ordinamento è incorso rispetto alla normativa comunitaria. Nel corso di questi anni, infatti, abbiamo sempre più appreso a concepire l'appartenenza all'Unione europea nella sua effettiva dimensione dinamica. L'Europa, quindi, non più e non solo un traguardo raggiunto una volta per tutte, ma una condizione che richiede di volta in volta di essere ridefinita e riadeguata in funzione degli ordinamenti vigenti, tanto il nostro quanto quello comunitario, che devono essere assunti come un *corpus* di norme vive che abbisognano di essere costantemente messe in fase e in sincronia tra loro. Tutti noi sappiamo che la disciplina in proposito è caratterizzata da una fase ascendente, di formazione delle direttive comunitarie, in cui i Parlamenti e i Governi degli Stati membri concorrono a vario titolo nella formazione delle direttive medesime, e da una fase discendente in cui invece gli stessi sono chiamati a recepire negli ordinamenti nazionali le disposizioni contenute nelle direttive. Come è stato ben evidente nel corso di tutti questi anni, assai più difficile e delicata risulta essere la seconda funzione rispetto alla prima. Di certo così è stato almeno per il nostro Paese, ritengo anche per il peso di un bicameralismo perfetto, quale il nostro, che mal si concilia rispetto ai tempi ed alle esigenze europee. Solo in tempi più recenti è stata giustamente adottata una decretazione d'urgenza per sanare proprio quelle procedure d'infrazione comunitaria che si trovavano ad un punto tale da incorrere nelle sanzioni previste, e comminate talvolta, dalla Corte di giustizia europea. In questo senso, lo strumento individuato è stato, ad ordinamento vigente, il più consono e di fatto quello che si è rivelato ad oggi il più efficace. Grazie a queste e ad altre misure è stato infatti possibile conseguire una sensibile riduzione del numero delle procedure di infrazione (lo ricordava la collega Bonino), che, per la prima volta dal 2002, è sceso - è bene ricordarlo ancora - al di sotto della soglia, anche psicologica, delle 200 infrazioni, con una riduzione complessiva di circa 80 unità nei soli due anni del precedente Governo. Il miglior risultato mai raggiunto dal nostro Paese!

Senza un immediato intervento legislativo che scongiurasse tale ricorso l'Italia rischiava per ciascuna delle procedure di infrazione contenute nel provvedimento la condanna al al pagamento di una somma forfetaria minima di circa 10 milioni di euro, oltre ad una penalità di mora compresa tra 22.000 e 700.000 euro per ogni giorno di ritardo nell'attuazione della seconda sentenza. Fin qui, potremmo dire, la doverosa ricostruzione dei fatti, che mi è sembrata, mi scusi il relatore, manchevole nella presentazione del provvedimento e che invece, anche per una nuova prassi istituzionale che inveri nella sostanza il riconoscimento delle azioni positive compiute nell'interesse del Paese, ritengo debba essere resa per amor di giustizia e ad onor del vero. Circa il merito del provvedimento, mi preme segnalare all'attenzione dell'Aula due aspetti, su cui anche gli interventi precedenti si sono concentrati, perché su questi non a caso, e certamente non per vezzo, abbiamo marcato la nostra azione e la nostra attenzione nel dibattito parlamentare, tanto alla Camera quanto oggi al Senato. Su di essi, come è evidente, non saremo disposti a fare sconti per il futuro. aspetti non marginali, non solo per la portata e il significato che gli emendamenti introdotti dal Governo assumono, ma anche per uno stile di comportamento che mal si concilia con una stagione nuova della politica italiana che tutti a parole vorremmo aprire, ma che voi, signori del Governo, sembrate per primi tradire nei fatti. Mi riferisco a quegli emendamenti che sono stati definiti nel dibattito alla Camera emendamenti «salva Retequattro» e «lodo Ermolli», con una qualche indubbia forzatura, senatore Grillo, ma anche - lasciatemelo dire, colleghi della maggioranza - con una qualche efficacia comunicativa che coglie bene un sentimento diffuso ai più nel Paese, un sentimento che ritengo a voi per primi non giovi alimentare per affrontare gli enormi problemi che questo Paese si trova davanti. questioni la cui attribuzione come eredità del Governo Prodi può magari tornare utile per vincere una campagna elettorale, ma non certo per risolvere problemi che invece vanno risolti davvero, come voi, cari colleghi, spero sappiate bene. Per intendersi, ciò vale tanto per Alitalia quanto per i rifiuti in Campania. altro rispetto avrebbero meritato le Aule parlamentari e le Commissioni di merito. Mi riferisco, come capite bene, in modo particolare all'emendamento non ritirato, e per termini di scadenza di fatto oggi blindato, che vedrà approvare *ex lege* le convenzioni alle concessionarie autostradali, saltando ancora una volta ogni controllo di merito degli organismi istituzionali preposti; alludo, come sappiamo, al parere del NARS, del CIPE e delle Commissioni parlamentari. Un atto questo tanto più grave per quanto l'intera vicenda ha assunto nel corso degli anni contorni di opacità e di singolare vischiosità. Un sistema che, come sappiamo, ha consentito nella gestione del processo di privatizzazione del sistema autostradale italiano, da un lato, l'attribuzione delle perdite al pubblico, in termini di mancati investimenti, e, dall'altro, la spartizione di lauti dividendi tra l'azionariato dei grandi gruppi privati e finanziari del Paese. Questa purtroppo è, in estrema sintesi, la travagliata e intricata vicenda, tutta italiana, del nostro sistema autostradale. Una situazione ancor più singolare in ragione del fatto che chiama in causa anche il mutevole ruolo dell'ANAS, che in questi anni doveva vigilare sull'effettivo interesse pubblico (costituito dalla resa degli investimenti e degli interventi che i concessionari dovevano effettuare), interesse che invece nel tempo è sembrato, per usare un eufemismo, rarefarsi. A queste sensazioni voi avete risposto con un *blitz*, che temo non vi comporterà neppure la riconoscenza dovuta. Un po' perché eccessiva è la posta che come contropartita chiedete, un po' perché questo è il nostro capitalismo. Lo dico senza disvalore per alcuno, ma come semplice constatazione nei confronti di imprenditori che nel tempo hanno assunto piuttosto la fisionomia dei «predatori di Stato», senza niente o poco (sicuramente troppo poco), dare in cambio. Ma allora, e concludo, a a chi giova questo provvedimento? A questa semplice e banalissima domanda, colleghi della maggioranza e rappresentanti del Governo, siete e sarete chiamati a rispondere al Paese. A questa semplicissima e banalissima domanda non potrete sottrarvi. A questa semplice e e banalissima domanda dovrete dare compiute e circostanziate risposte per un operato che fino ad oggi non ha certo brillato per trasparenza ed efficacia. Allora, in ultimo, una sola raccomandazione: una volta tanto, se possibile, queste risposte datele senza facili slogan o simpatici mottetti.

molti si sono allargati a tematiche particolari: a me, in chiusura di questo dibattito, piace ricondurre il tutto al tema di fondo, che è quello di un adempimento non solo formale né secondario. Siamo chiamati, ad un adempimento di vitale importanza per i rapporti tra l'Italia e l'Unione europea: la trasposizione in legge del decreto-legge sugli obblighi comunitari

II provvedimento riveste caratteri di particolare necessità ed urgenza anche per l'evento imprevisto, fino a qualche mese fa, delle elezioni anticipate. Parte del lavoro infatti fu svolto dal Governo morente, altra parte da quello nascente. Quindi, c'è stato un momento di vuoto che certamente non ha giovato alla trasparenza. II passaggio, dicevo, non è rituale ma sostanziale. Le disposizioni che ci apprestiamo a votare hanno come scopo quello di scongiurare il deferimento dell'Italia alla Corte di giustizia ed evitare che le procedure di infrazione procedano nelle loro fasi, fino a quella ultima, più grave, sanzionatoria. Come ha ben detto - anzi, mi complimento con lui - il relatore Malan, un'eventuale condanna dello Stato italiano per inottemperanza al giudicato comunitario nelle infrazioni così considerate porterebbe al pagamento di una multa di quasi 10 milioni di euro, oltre ad ulteriori aggravi

è che il lavoro su questo terreno finisca qui: sappiamo che rimangono aperte a carico dell'Italia circa altre 200 procedure di infrazione e quindi non possiamo certo permetterci di abbassare la guardia. Ma non sia quello di oggi, signor Presidente, signori membri del Governo, signor relatore, solo solo un atto dovuto, quasi notarile, formale. Noi oggi abbiamo anche la possibilità di alzare un po' l'orizzonte, di ribadire i buoni motivi per i quali da sessant'anni l'Italia è Paese fondatore e convinto sostenitore del sodalizio europeo e della sua sempre maggiore attualità, nonostante un crescente scetticismo da parte anche di alcune componenti italiane del Parlamento. Non solo, ma abbiamo anche l'opportunità di confermare, attraverso linee programmatiche e ideali politici, il modo in cui noi italiani intendiamo stare in Europa, nel grande concerto dei 27 Paesi membri, alcuni dei quali fondatori, quindi consolidati, altri di successiva (alcuni addirittura recentissima) acquisizione. E su come noi stiamo in Europa ci stanno guardando in molti. Essere in regola con i conti impegnarsi per il recupero del debito pubblico, attraverso il controllo del deficit*,* è sicuramente il segnale più convincente del nostro stile, della nostra convinzione di essere parte attiva, parte soprattutto viva del concerto europeo, ma è anche il modo più concreto per essere credibili ed autorevoli nelle decisioni che contano. Un Paese che rispetta le regole è un Paese più ascoltato ed apprezzato, nonché più sostenuto nelle battaglie assembleari, dal Parlamento europeo al Consiglio europeo. È lapalissiano come tutto questo possa tradursi, in termini di consenso, anche in maggiori opportunità nel trasporre interessi nazionali, linee italiane, nella produzione legislativa comunitaria. Oggi più che mai abbiamo bisogno di questo consenso e di questa stima diffusa nel momento in cui problemi apparentemente italiani, come per esempio quello dell'immigrazione, debbono viceversa diventare tematiche generali, tematiche europee allargate e condivise da tutti i Paesi membri, ciascuno dei quali deve farsene carico. Non è quindi solo un problema di uno Stato, ma di tutta la società europea. Eccellenti risultati in questo senso sono scaturiti dalle prime uscite pubbliche dei rappresentanti del nuovo Governo nei vari consigli tecnici a Bruxelles. È di questo inizio di settimana (ieri o l'altro ieri) la promozione dell'Italia e del ministro Tremonti nel corso di una riunione dei Ministri economici a Francoforte, dove si è celebrato il primo decennale di vita della Banca centrale europea. La relazione, molto coraggiosa, del nostro Ministro è stata a lungo applaudita e i suoi punti salienti, come l'abolizione dell'ICI, la detassazione degli straordinari e i provvedimenti sui mutui, che nel nostro Paese sono stato accolti in maniera variegata, sono stati viceversa accettati e commentati come novità stimolanti, da alcuni Paesi perfino indicati come esempi da poter applicare e seguire. Jean-Claude Juncker, un un presidente molto arcigno dell'Eurogruppo, ha detto esplicitamente che il piano italiano va bene per quello che sana per il passato e per quanto prevede per il futuro. Anche il commissario Almunia, che è solitamente piuttosto arcigno verso l'Italia, ha detto che siamo sulla strada giusta. Il ministro Tremonti ha confermato il percorso che ci consentirà di rientrare dal deficit e di raggiungere il pareggio dei conti nel 2011, un anno prima della della Francia, che ha chiesto la proroga al 2012. Questo è un altro passo importante per il recupero da parte dell'Italia del ruolo di Paese guida, di Paese modello che aveva perduto negli ultimissimi tempi. Ora il nostro impegno deve sapersi trasferire anche sul terreno più istituzionale, per esempio quello della ratifica del Trattato di Lisbona, un documento deludente se pensiamo alla splendida

abbandonata sotto la spinta degli euroscettici. Il Trattato di Lisbona ne ha recuperato sicuramente le linee fondamentali, ma quel respiro e quello slancio di allora, che avrebbero portato l'Europa al grande balzo verso le comuni istituzioni politiche, vanno mantenuti come estrema speranza, come obiettivo per un'Unione che forse domani sarà più pronta e matura per recepire tutto questo. Ora anche l'Italia deve ratificare il Trattato di Lisbona e l'appello che mi sento di rivolgere è di farlo per vie parlamentari, come hanno fatto altri 12 Stati membri, compresi alcuni di recente acquisizione. Anche l'area dell'euro si va allargando, segno che la consapevolezza che l'unione monetaria è la sola via per favorire la crescita, lo sviluppo e la stabilità sta raccogliendo consensi anche in Paesi una volta scettici. Il 1° gennaio arriverà la Slovacchia e così l'euro conterà 16 Paesi. Proprio in questi giorni la antica, la romantica politica agricola, la madre di tutte le politiche europee, ha varato l'ennesima coraggiosa riforma per mantenersi al passo con i tempi e con le mutate regole del mercato. Infine, l'Unione europea sta spingendo sull'acceleratore di quella che viene definita l'Europa dei cittadini. L'Unione europea vuole essere sempre più un'area aperta, favorire una convinta partecipazione della gente ai programmi comunitari e alle iniziative di democrazia diffusa. Da Maastricht in poi, è chiaro a tutti, non di solo mercato vive l'Europa ma, signor Presidente, signori colleghi, nemmeno di polemiche sulle frequenze televisive.

il sottosegretario Romani, che saprà con grande abilità e competenza replicare a tutte le critiche sollevate su questo terreno. In chiusura, signor Presidente, annuncio che il Popolo della Libertà voterà a favore di questo provvedimento, ma non come un atto dovuto, bensì come conferma della nostra incrollabile vocazione europeistica.

il senatore Formigoni dichiara di dimettersi dalla carica di senatore, al fine di proseguire il proprio mandato di Presidente della Regione Lombardia. Trattandosi di dimissioni motivate da incompatibilità ai sensi dell'articolo 122 della Costituzione, l'Assemblea non può che prenderne atto. La Giunta delle elezioni è autorizzata a convocarsi, ai fini dell'individuazione del senatore subentrante, che sarà proclamato all'inizio della seduta pomeridiana. **Su *(LNP)*. Signor Presidente, mi scusi, vorrei fare presente all'Assemblea un gravissimo episodio verificatosi questa mattina a Mestre (Venezia) contro una nostra sede. 70 no global sono entrati nella sede della Lega Nord di Mestre, malmenando un nostro militante, pensionato, che la custodiva, buttando all'aria l'arredamento e impossessandosi di nostre attrezzature. A capo di questo commando di violenti picchiatori del centro Rivolta c'è tal Tommaso Cacciari, rampollo della famiglia del sindaco di Venezia, evidentemente indispettito perché il nostro movimento, con gli amici del Popolo della Libertà, si sta opponendo alla costruzione di un campo nomadi in quel di Mestre, in una zona fortemente urbanizzata, che costerebbe 3 milioni di euro, sottratti alle necessità primarie dei veneziani. Le chiedo, signor Presidente, a nome del Gruppo della Lega Nord, un intervento in Aula del Ministro dell'interno, per fare chiarezza su questo gravissimo atto antidemocratico contro esponenti e strutture del nostro movimento